un anno fa, una gravissima esplosione seminava morte e distruzione intorno alla stazione ferroviaria della città di Viareggio. Nel breve volgere di pochi istanti, le fiamme sprigionate dal deragliamento di un convoglio ferroviario carico di gas inghiottirono le case e le strade accanto ai binari, provocando la morte di 32 persone, tra le quali purtroppo si contarono diversi bambini e ragazzi. Alcune delle vittime - è terribile ricordarlo - perirono dopo settimane o mesi di indicibili sofferenze per le ustioni subite. Come ho ricordato oggi in un messaggio inviato al sindaco di Viareggio, questa assurda tragedia poteva essere evitata. Al di là delle responsabilità penali, che è compito della magistratura accertare e far valere, è fuori di dubbio che una più solida cultura della sicurezza, basata su un'applicazione ferma e rigorosa delle norme vigenti, ed un governo del territorio che consideri anche i rischi potenziali per la salute e la sicurezza dei cittadini, divengono la condizione indispensabile perché una vicenda come questa non abbia mai più a ripetersi. Nelle scorse settimane, nell'incontrare i familiari delle vittime dell'esplosione, ho manifestato loro la ferma volontà delle Istituzioni parlamentari di accompagnare e sostenere il loro doloroso, quotidiano cammino verso la riconquista della normalità. Credo che l'approvazione definitiva in sede deliberante, con voto unanime di tutte le forze politiche, di un disegno di legge che mette a disposizione delle famiglie delle vittime e di tutti quanti hanno riportato gravi lesioni un fondo di 10 milioni di euro, avvenuta cinque giorni or sono da parte della Commissione lavori pubblici del Senato, costituisca il segno più tangibile della fattiva volontà del Parlamento di non lasciare soli quanti hanno subito nel corpo e nei legami familiari i terribili effetti di quella strage. Invito allora tutti i colleghi ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento, nel commosso ricordo delle 32 vittime della tragedia di Viareggio.

ad un anno dalla strage di Viareggio, oggi ancora non conosciamo le vere responsabilità, ma ci interessa e ci appartiene, nella cultura del rispetto, da parte del nostro Gruppo esprimere la piena solidarietà, la piena condivisione per il dramma che ha colpito le famiglie dei 32 cittadini scomparsi. Abbiamo cercato di fare il nostro dovere in 8a Commissione e credo che - proprio come è stato ricordato in sede deliberante - sia stato raggiunto l'obiettivo di fondo:

Gruppo: fino a che punto il profitto sarà in grado di togliere speranza e sicurezza nella vita? Dico questo perché sono state compiute audizioni, incontri analisi sulle responsabilità. Credo che tale monito possa costituire prospettiva per il futuro nel momento in cui

Signor Presidente, anche noi ci associamo alle parole che lei ha voluto formulare a distanza di un anno dalla tragedia di Viareggio. Ci associamo altresì al dolore della città dei familiari delle 32 vittime. Condividiamo ed apprezziamo quanto il Senato e l'8a Commissione permanente hanno fatto come prima risposta, primo gesto di vicinanza e di solidarietà delle istituzioni nei confronti di chi è stato colpito da questa tragedia. È in corso un'indagine della magistratura che, ovviamente, cammina su un binario - diciamo così - parallelo rispetto

che hanno prodotto questo tipo di evento, capire se le nostre stazioni - la stragrande maggioranza delle stazioni ferroviarie che attraversano il cuore delle città

Signor Presidente, onorevoli senatori, ricordiamo con dolore la tragedia di Viareggio, che ha colpito la sensibilità dei cittadini per le sue modalità, per quelle fiamme nella notte che richiamavano l'inferno, per lo strazio le vite umane bruciate in un attimo, per una responsabilità oggettiva. Ancora si indaga, ma - come spesso accade nel nostro Paese le vittime e i loro familiari non riescono ad essere né risarciti né riscattati. Si deve allora dare atto a questa maggioranza e a tutto il Parlamento che, di fronte all'emergenza, si sanno muovere con tempestività, efficacia e concretezza. Si è intervenuti in modo significativo con ragionevole rapidità rapidità e proprio qui al Senato, come ha ricordato lei, signor Presidente, siamo già in una fase avanzata di quel processo che deve portare sollievo in tutti i sensi a chi è stato colpito. il caso - e me ne guardo bene - di assumere toni retorici e tanto meno trionfalistici. Mi pare, però, si possa ascrivere a questo Parlamento il merito di non trasformare il terremoto dell'Aquila in un'altra Irpinia e la tragedia di Viareggio in un dramma suggellato dai telegrammi di cordoglio della prima ora. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorre il primo anniversario del disastro ferroviario che ha sconvolto Viareggio, che ha causato la morte di 32 persone e centinaia di feriti. Il 29 giugno del 2009, poco prima di mezzanotte, un treno merci transita dalla stazione di Viareggio: procede da nord verso sud, da La Spezia in direzione di Pisa, col suo convoglio di 14 vagoni cisterna carichi gas. La stazione è stata appena superata quando il treno raggiunge una linea ferrata costeggiata dai palazzi; in parallelo corre via Ponchielli. È in questo punto che il merci 50325 deraglia. Il primo carro cisterna trascina fuori dai binari altri quattro dei 14 vagoni che non sono proprietà delle Ferrovie dello Stato, ma appartengono a una società straniera, la Gatx con sede a Vienna. Solo uno si spezza, urtando contro un paletto di ferro piantato in prossimità dei binari: purtroppo basta a causare l'immane disastro. Le esplosioni e le fiamme investono i palazzi e la strada. Una palazzina, dove vivono 18 persone, si sbriciola. Una più piccola, monofamiliare, prende fuoco. A pochi minuti dalla mezzanotte, via Ponchielli non esiste più. I segnali premonitori erano stati numerosi sulla rete ferroviaria; nessuno, tuttavia, decise di intervenire. Le responsabilità debbono, dunque, essere accertate. La giustizia sta facendo il suo corso e noi, con fiducia nella magistratura, aspettiamo. È un dolore grande per tutta la città, e una responsabilità enorme per tutte le istituzioni. Quest'Aula ha onorato il proprio ruolo, proprio pochi giorni fa, grazie all'impegno straordinario del presidente Schifani e con la collaborazione di tutti i colleghi, nessuno escluso, approvando una legge straordinaria che prevede un risarcimento di 10 milioni milioni di euro per i familiari delle vittime. Un ringraziamento particolare va al relatore, il senatore Baldini, e alla senatrice Granaiola La Regione Toscana, attraverso il commissario Martini, a cui è subentrato il nuovo presidente Enrico Rossi, ha già speso 15 dei 19 milioni di euro per la ricostruzione. Ma ad un anno da quel disastro dobbiamo assumere l'impegno politico e morale di rendere il trasporto delle merci pericolose più sicuro. pochi mesi dopo la tragedia di Viareggio lo stesso treno merci ha preso fuoco a Giuncarico, nei pressi di Grosseto, trasportando nuovamente GPL, e questo è un pericolo che ancora esiste sulla nostra rete. Dobbiamo fare una verifica a tutto campo, non solo per i cittadini di Viareggio, ma per tutto il Paese. Interpretando il sentimento di tutto il Senato, voglio esprimere a nome del Gruppo del Partito Democratico il mio cordoglio ai familiari delle vittime ed alla città di Viareggio per questo triste, drammatico primo anniversario della strage, con l'impegno di tutti perché episodi come questo non accadano più. il Gruppo del Popolo della Libertà si associa commosso alle espressioni di cordoglio che hanno contraddistinto Il ricordo della vampa di fuoco che incendiò l'aria, vaporizzando tutto ciò che trovava al suo passaggio in un abbraccio mortale che travolse sia i nostri connazionali, sia quanti in questo Paese erano venuti alla ricerca di miglior sorte, è ormai indelebilmente impresso nella memoria collettiva di ciascuno di noi. Ed è toccante e significativo che proprio oggi l'unica sopravvissuta di una famiglia che da anni viveva nel nostro Paese abbia ricevuto la cittadinanza italiana grazie a un decreto del Presidente della Repubblica, che ha voluto dedicare parole particolarmente commosse a questo tragico evento. È giusto sicuramente rispettare la volontà espressa dai familiari delle vittime di stringersi oggi intorno solo al primo cittadino di Viareggio, quasi a chiedere alla politica ed alle istituzioni di fare un passo indietro. Però, al di là di ogni strumentalizzazione, è giusto e doveroso ricordare che, forse, in questa vicenda tragica più che in altre, la politica e le istituzioni, il Parlamento in particolare, hanno saputo mostrarsi all'altezza della situazione. L'opera di ricostruzione è già significativamente avanzata. Il Parlamento ha adottato provvedimenti che vanno nella direzione di assicurare l'unica possibile forma di risarcimento - ahimè! - nei confronti delle vittime, sono stati presi significativi provvedimenti per il potenziamento della sicurezza. Infatti, se noi vogliamo onorare fino in fondo la memoria di quelle vittime, dobbiamo far sì che quella cultura della sicurezza alla quale ella, signor Presidente, sia sempre costantemente oggetto di particolare tutela e presidio da parte di ciascuno di noi. riunitasi il 25 giugno scorso, ha preso atto a maggioranza della necessità - posta dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento - di convocare l'odierna seduta straordinaria dell'Assemblea per la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di spettacolo e attività culturali, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in scadenza nella giornata di oggi. I tempi sono stati ripartiti in ragione di 20 minuti per ciascun Gruppo, comprensivi anche delle dichiarazioni di voto, affinché il voto finale possa avere luogo entro le ore 18,30 e consentire, quindi, la promulgazione del provvedimento nel termine costituzionale. A tal fine, come già preannunciato ai Capigruppo, la Presidenza - ove si rendesse necessario in relazione all'andamento dei lavori - potrà avvalersi degli strumenti offerti dal Regolamento per assicurare la votazione finale del decreto, che scade in data odierna, entro il termine predetto. Inoltre, nel prendere atto della richiesta unanime della 5ª Commissione permanente di poter disporre di tutta la settimana corrente per completare l'esame del decreto-legge sulla manovra economica, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di fissare per la seduta pomeridiana di martedì 6 luglio l'avvio della discussione del provvedimento. Pertanto le sedute dell'Assemblea già previste per giovedì 1° e venerdì 2 luglio non avranno luogo, mentre resta confermata la convocazione del Parlamento in seduta comune giovedì 1° luglio, alle ore 9, per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. In relazione alla richiesta della Commissione bilancio, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge relativo alla manovra economica è stabilito per le ore 14 di lunedì 5 luglio. Prima dell'inizio della seduta pomeridiana di martedì 6 luglio, sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire - anche in relazione al numero di emendamenti presentati - la ripartizione dei tempi tra i Gruppi e la complessiva organizzazione dei lavori per la discussione del provvedimento. In relazione alla richiesta del Gruppo UdC-Autonomie di una sollecita iscrizione nel calendario dei lavori del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la Presidenza ha invitato i Presidenti delle Commissioni competenti ad organizzare i propri lavori al fine di consentire un prossimo esame da parte dell'Assemblea. In una delle prossime sedute sarà ricordata la figura di Pietro Milio, nonché, come richiesto dalla senatrice Finocchiaro a nome del proprio Gruppo, di Rina Gagliardi, già componenti del Senato in precedenti legislature, recentemente scomparsi. Presidente, rubo poco tempo alla discussione e al nostro impegno per terminare entro l'ora prevista. È un impegno che intendiamo rispettare, ma ci sono due questioni delle quali vorrei parlare. La prima riguarda

temo di vedere - mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza - uno straordinario scarto tra quello che sui giornali è l'interesse che nel Paese e in molte delle sue istituzioni è

sui cittadini italiani e, in particolare, sui cittadini più esposti anche sotto il profilo soltanto del loro reddito. Di fronte a tutto questo, potremmo dire che in

proprio lavoro), nella difficile situazione di chi, appunto, non può dir parola, non ha una parola da poter spendere e che attende che si compensino altrove, in altri luoghi e non in Parlamento, gli interessi che devono essere compensati perché alla maggioranza arrivi l'ordine.

né la partecipazione, né la proposta, né la discussione; ma lo dico anche perché forse è bene che si sappia anche fuori da qui - ammesso che queste mie parole abbiano un'eco, perché non so se c'è la se c'è la notizia, come si dice in gergo - che mentre il Paese si interroga - e con quale forza, con quale mobilitazione, con quale pienezza di argomenti! - su questa manovra finanziaria, nella Commissione bilancio del Senato c'è la simulazione di una discussione, una recita a soggetto in cui peraltro il copione non è scritto neanche dalla maggioranza parlamentare, ma è scritto altrove e verrà poi calato, e su questo i colleghi della maggioranza si acconceranno a recitare e i colleghi dell'opposizione si acconceranno a fare il loro lavoro. Quanto questo giovi al Parlamento, all'esercizio della funzione parlamentare e al Paese e, mi si lasci dire, anche alla maggioranza e al Governo, francamente non riesco a vederlo.

Prima della sua convocazione, la Conferenza dei Capigruppo da lei presieduta aveva convocato l'Assemblea per il 1° luglio. Dopodiché, la modificazione che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, l'ha indotta ad una convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento. Vorrei richiamare a lei e all'Assemblea anche il disposto dell'articolo 56, comma che riguarda l'ordine del giorno della seduta. Esso dispone: «Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta».

assuma un po' le funzioni delle sezioni unite della Corte di cassazione e, quindi, metta un punto fermo. Infatti, la convocazione dell'Assemblea del Senato

anche quando non è prevista alcuna seduta in calendario e se anche quando vi è mancato accordo tra i Presidenti dei Gruppi

Per questo chiedo di non aprire la discussione senza aver prima convocato la Giunta per il Regolamento,

ognuno di noi sia in condizione di andarli a guardare sul sito del Senato per averne contezza prima di venirne a discutere, e in Conferenza dei Capigruppo e, eventualmente, nell'Aula del Senato. apre una nuova finestra"). Senatore Belisario, lei osserva che la decisione di modificare il calendario dei lavori del Senato per inserirvi la seduta odierna sarebbe stata adottata dalla Conferenza dei Capigruppo con il voto contrario del rappresentante dell'Italia dei Valori, il che risponde a verità. Ma come ho già rilevato nella Conferenza dei Capigruppo di quel venerdì 25 giugno, a norma dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, il Presidente del Senato ha un autonomo potere di modificare il calendario «per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso». Questo è appunto il caso di specie, in cui il calendario è stato modificato per consentire al Senato di esaminare il disegno di legge di conversione di un decreto-legge in scadenza. Conformemente alla prassi, pur trattandosi nella fattispecie di esercitare un potere di competenza del Presidente del Senato, la Conferenza dei Capigruppo è stata convocata, sia come gesto di cortesia e di rispetto nei confronti dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sia per giungere ad una organizzazione condivisa della discussione. condivisa della discussione. Il termine in questione, secondo la Presidenza e tutti i precedenti, ha carattere ordinatorio e non vincolante. Il citato comma 1 dell'articolo 56 infatti prescrive che nei casi di convocazione a domicilio, quale è il caso in specie, la diramazione dell'ordine del giorno è fatta «di regola» almeno cinque giorni prima della seduta. In definitiva, il termine di cinque giorni può essere derogato quando le circostanze lo richiedano. Così è nel caso presente, poiché la seduta odierna è stata convocata nell'ultimo giorno utile per consentire al Senato di esaminare il disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Numerosi precedenti, inoltre, confermano che la disposizione dell'articolo 56, comma 1, è costantemente interpretata nel senso ora detto, tanto che, se necessario, la convocazione straordinaria è stata disposta persino un giorno per quello successivo a quello in cui veniva disposta, cioè con la distanza di un solo giorno. Gli Uffici, senatore Belisario, sono a disposizione della sua persona e degli onorevoli senatori per fornire nel dettaglio tutti i precedenti relativi.

Vi erano iscritti altri senatori, ma non si è potuto procedere in tal senso. Quindi, ci presentiamo in Aula, signor Presidente, senza aver approvato un testo e senza aver dato nessun mandato al relatore, senatore Asciutti.

Signor Presidente, abbiamo rinnovato la questione pregiudiziale dopo che il testo è tornato dalla Camera, come avevamo già fatto nella prima lettura qui al Senato, perché speriamo che anche la maggioranza possa avere modo di ripensare ai profili di incostituzionalità che abbiamo sollevato con tale questione.

ben poco, o nulla, hanno a che vedere con la decretazione d'urgenza. Il presidente Napolitano, abbastanza recentemente, ha richiamato tutti i parlamentari

Questo è proprio il caso del decreto sugli enti lirici. È un gran pasticcio. Oggi in Commissione, prima dei lavori sono stati fatti anche degli appunti da parte della maggioranza rispetto alle modifiche introdotte frettolosamente alla Camera. E la stessa maggioranza si è interrogata sul significato di queste modifiche che sono state introdotte. E questo purtroppo è il risultato della fretta nell'esaminare un provvedimento che avrebbe invece richiesto i suoi dovuti tempi, la sua dovuta e importante discussione e il suo dovuto confronto. Fra l'altro, questo è un tema su cui i lavori della Commissione al Senato avevano già prodotto importanti risultati. Era stata approvata anche una risoluzione che vedeva fra l'altro, come primo firmatario, il nostro capogruppo in Commissione, era stata anche cofirmata dal rappresentante della Lega Nord. Quindi era un lavoro importante di confronto quello che era stato fatto, e che avrebbe potuto sfociare in un disegno di legge ordinario che avrebbe consentito in Commissione ed in Aula una discussione importante, pacata ma sicuramente più fruttuosa di quella fatta con la decretazione d'urgenza.

questa maggioranza e il Governo Berlusconi privino il Senato, la Camera e quindi le Aule parlamentari di una discussione serena e importante che ci sarebbe potuta essere. Grazie, Presidente. il testo che oggi è qui per la terza lettura, ancorché sia stato arato da qualche emendamento nel corso del viaggio tra il Senato e la Camera, rimane profondamente inaccettabile e certamente viziato da evidenti profili di illegittimità costituzionale.

secondo i termini discussi più di un anno fa in Commissione 7a, non ha nulla a che fare con i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, che anzi in questo caso davvero sono aggirati in modo clamoroso. Non c'era infatti alcuna urgenza,

che l'articolo 117 della Costituzione assegna alle Regioni un ruolo molto specifico e la riforma del Titolo V della Costituzione aveva dato specificamente proprio alle Regioni una fisionomia del tutto diversa da quella che si evince dall'articolato del decreto-legge.

dei rapporti tra Stato e Regioni. Si può supporre - faccio una facile previsione - che qualche Regione ricorrerà e il fragile testo che si sta per discutere

invece vengono con dirigismo autoritativo calpestate nella loro fisionomia. Ecco un altro argomento che andrebbe considerato, se si vuole prestare orecchio, nel valutare questa normativa incostituzionale. Insomma, è un testo inaccettabile e lo dico anche perché fa il paio con tanti tagli in corso d'opera alle attività culturali, alle attività dei saperi, alle attività dell'informazione, insomma

e colga le preoccupazioni che noi poniamo. Perché noi vorremmo una riforma, noi vorremmo che finalmente il settore si dotasse di una legislazione moderna, evoluta e adatta al secolo della conoscenza e della multimedialità. Così non è: questo decreto ci riporta indietro, toglie anche quel poco di bello che c'era nella normativa pregressa, la rende forse inapplicabile e anche per questo esso davvero non ha senso ed a poco valgono alcuni ritocchi se il contesto è rimasto e rimane quello. Ecco perché invito le colleghe e i colleghi a votare per questa nostra pregiudiziale, che non è un pre‑giudizio: è invece un giudizio su un articolato nel senso

a richiamare un aspetto di questo provvedimento che già nei lavori della Commissione ho evidenziato. Il mondo della cultura, in particolare il mondo delle fondazioni lirico-sinfoniche, come tutti

che si è voluto fare in fretta e furia sostanzialmente la montagna ha partorito il topolino. Siamo partiti da un testo che era molto aulico nel titolo, dove si parlava di riforma dell'ordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma che di riforma,

per fare quel che vorrà, senza una larga discussione e una partecipazione da parte del mondo della cultura nel suo complesso, e quindi è l'ennesima imposizione da parte del Governo Berlusconi. [**Presidenza della vice presidente

come se i costi di uno spettacolo fossero da addebitarsi esclusivamente agli artisti e alle maestranze. Ciò è stato mortificante.

In uno degli emendamenti approvati alla Camera si è avuto persino il pudore di sopprimere le parole iniziali del secondo articolo, in cui si diceva «in attesa della riforma», perché, forse, i nostri colleghi della Camera erano consapevoli che, giunti a questa fine, alla fine dell'esame del decreto-legge e degli enti lirici, non ci sarà più riforma. Molti dei 14 enti correranno il rischio di chiudere i battenti se non troveranno sui loro territori, nonostante i tagli agli enti locali, aiuto da parte dell'associazionismo culturale, da parte delle fondazioni bancarie, da parte dei Comuni.

di godere di uno spettacolo bellissimo all'Arena di Verona. È stata un'esperienza per molti ripetuta, ma che serve a ricordare che cosa significa il Festival di Verona. È una fondazione, dal punto di vista giuridico,

alcuni incentivi a questi professori d'orchestra significa non conoscere bene la loro professione, né i risultati artistici che ottengono a favore dell'intera cultura italiana e dell'indotto dal punto di vista turistico, né il costo

mentre voi, come maggioranza e Governo, ottenete uno strumento che serve solo a contenere e ad ulteriormente ridimensionare i costi. Non so quando avremo una riforma che serve all'intero Paese. Vorrei rappresentarle, signor Ministro, la nostra sorpresa, il rammarico di chi anche in politica pensa che mantenere la parola significa trovare gli strumenti per realizzare gli obiettivi comuni.

Ci sono altri emendamenti ancora più puntuali, perché oggi, signor Ministro, pur sapendo che sarebbe stato limitatissimo il tempo in Commissione e limitato il tempo in Aula, non avevamo nessuna intenzione

la vera industria immateriale dell'Italia. Un Paese senza materie prime può investire esattamente nei saperi,

dei tesori più preziosi che il nostro Paese mette a disposizione non solo degli italiani, ma del mondo intero. Signor Ministro, colleghi, credo che amputare parti importanti di cultura significhi rendere meno vivo il Paese e non elevare culturalmente anche le persone modeste. Lei, signor Ministro, saprà che tra i melomani ci sono molte persone che non sono di grande cultura;

il riconoscimento del valore manageriale del sovrintendente, che avrà responsabilità diretta. Tale emendamento è stato accolto alla Camera, e noi lo riconosciamo come utile, ma riconosciamo anche che probabilmente in futuro potrà godere di questa magnifica arte solo chi potrà pagare il biglietto: gran parte dei melomani non potranno farlo, a causa del fatto che i sovrintendenti dovranno recuperare soldi anche attraverso la biglietteria. Non potranno più goderne, ed è un rimpianto aggiuntivo. *(Applausi dai Gruppi

Signora Presidente, onorevoli senatori, mi dispiace che alcuni colleghi dell'opposizione, riprendendo il dibattito che si è svolto in quest'Aula pochi giorni fa, abbiano parlato, riguardo al provvedimento sulle fondazioni lirico-sinfoniche, di un pasticcio e non invece di un fatto nuovo e positivo avvenuto nel nostro Paese e nel Parlamento. Mi sarei aspettato francamente che, oltre a ribadire da parte dell'opposizione un giudizio negativo del provvedimento che il Governo ha presentato, si tenesse conto anche delle novità positive che vi sono state nel corso del dibattito parlamentare; un dibattito che, come ho ricordato

si è svolto in maniera seria, responsabile e costruttiva fra le forze politiche, fra la maggioranza e l'opposizione, e che ha consentito

il dibattito e il confronto che si è svolto in quest'Aula, e soprattutto dopo il dibattito e il confronto che si è svolto alla Camera dei deputati,

con profonde modifiche al decreto sulle fondazioni lirico-sinfoniche, mi sarei aspettato, soprattutto da parte del Partito Democratico, delle parole diverse da quelle che ho ascoltato oggi. Mi sarei aspettato soprattutto che il Partito Democratico rivendicasse i propri meriti nell'aver anche ottenuto delle modifiche, delle integrazioni, dei miglioramenti al decreto-legge che stiamo discutendo. Questo vuol dire allora che il confronto è inutile, che il ruolo del Parlamento è inutile, che è inutile cercare il confronto tra le forze politiche, aprire il confronto tra le forze politiche, offrendo la disponibilità a profondi cambiamenti di un provvedimento di legge? Vuol forse dire che la fiducia è l'unica forma di decisione possibile in questo Paese? Io non lo credo; continuo a non a non ritenerlo e continuo a pensare che sia stato giusto impostare così il confronto e la discussione. Sono convinto che il decreto-legge che oggi spero il Senato approverà in via definitiva sia un provvedimento migliore di quello che il Governo ha presentato in Parlamento sono soddisfatto per una riforma che era necessaria e che pone le condizioni davvero - oggi sì - di un rilancio su basi nuove dell'opera lirica nel nostro Paese.

Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

forte, ossia: «Riforma! Riforma!». Il Partito Democratico, ma - devo dire - tutti i membri della 7a Commissione del Senato hanno richiesto con grande forza e grande foga la riforma degli enti lirico-sinfonici. Il Paese, i teatri d'opera, il mondo della lirica e della musica tutto, la cultura e i suoi protagonisti vogliono far vivere questo immenso patrimonio: la musica lirico-sinfonica. Vedete, il mondo ci guarda; ci guarda, ma non capisce, non può capire. Rimarrà scritto nelle peggiori pagine della politica il modo, la determinazione, l'inconcludente decisionismo, la mancanza di visione politica rispetto alla cultura, la volontà di umiliazione di un patrimonio fatto di storia, di grandi compositori, di grande tradizione e passione, ma anche di professionalità, di artisti, di maestranze che ci sono invidiate da tutti i grandi teatri del mondo.

Meglio, dove deve portare gli enti lirico-sinfonici? Bene, signor Ministro, non ci porterà da nessuna parte: ci porterà verso il niente. Con la risoluzione del marzo 2009 tutte le forze politiche erano pronte ad approvare una vera riforma nell'interesse della musica lirico-sinfonica, nell'interesse della nostra cultura, nell'interesse soprattutto del nostro Paese. Il Governo ha preteso una delega in bianco. Il Parlamento non può concedergliela, viste le reali volontà evidenziatesi in questo dibattito. Signor Ministro,

Occorre fare alcune considerazioni - pochissime - sull'ordine del giorno in esame. Questo ordine del giorno racchiude il lavoro importante che abbiamo svolto in 7a Commissione - lo ricorderà bene, signor Ministro - dove avevamo individuato le linee guida di una vera riforma

in terza lettura e che mortifica i tanti lavoratori del mondo dello spettacolo. Noi voteremo a favore di questo ordine del giorno perché riafferma che quel percorso che avevamo individuato in Commissione era quello giusto, e non a caso voi oggi ci date il parere contrario.

Perché nella precedente circostanza nella quale abbiamo discusso di questo provvedimento, tutti gli emendamenti poi recepiti alla Camera furono respinti? Signora Presidente - la prego di estendere questa mia considerazione al presidente Schifani - quando abbiamo approvato la legge sulle intercettazioni, è stato detto che finalmente era stato raggiunto un equilibrio intangibile, inalterabile, inossidabile. Dal giorno dopo la Camera dei deputati ha iniziato a ridiscutere il tutto,

la Camera lo ha messo radicalmente in discussione. Il mio quesito riguarda in cosa dovrebbe consistere il bicameralismo in Italia: che vi sia un ramo del Parlamento che prende atto delle modifiche che vengono apportate nell'altro ramo? E in che modo la maggioranza si rende disponibile a operare delle modifiche che non siano semplicemente la ratifica delle modifiche apportate alla Camera dei deputati? questo sia un tema di riflessione che attiene certamente alla dignità e alla utilità del nostro lavoro collegiale, all'efficacia del contributo dell'opposizione, ma anche, se posso dirlo,

discussione e un saggio confronto tra maggioranza e opposizione, e l'altro ramo in cui si viene in Aula soltanto per dire sì o no ad un testo manipolato nell'ambito di un accordo interno alla maggioranza, a quel punto qualcuno ci deve spiegare perché debba esistere

economici, che impoveriscono le risorse, e le intenzioni neocentraliste, che impongono direttive imperiose e tolgono autonomia, a fronte di una situazione di rivolta pubblica che richiede, invece, una maggiore concessione di risorse da destinare ad un settore in cui la cultura italiana è considerata giustamente, anche se forse certe volte con una certa generosità, all'avanguardia.

che lamentano l'impoverimento che deriverebbe da questo provvedimento, chiedendo invece il rispetto

consapevoli che all'interno del provvedimento al nostro esame ciò che domina è piuttosto l'idea della commercializzazione stretta e la ricerca di una sottrazione di autonomia analoga a quella ravvisabile nel provvedimento sulla scuola e sull'università. Torneremo su questo punto anche in occasione dell'esame di altri emendamenti.

prevede che, dopo le parole «alla designazione», vengano inserite le seguenti: «per tramite di dettagliati elenchi redatti dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti delle fondazioni». fondazioni». Tali elenchi, tra cui bisogna scegliere, sono quelli relativi ai membri del consiglio di amministrazione delle fondazioni e ai sovrintendenti. Non ho altro da

che ha ritenuto giusto intervenire sull'emendamento 1.23, avrebbe dovuto essere più

nell'Aula del Senato dica che non va bene e poi nell'Aula della Camera dica il contrario. Questo è il punto politico che il collega Rutelli voleva porre all'attenzione di tutti noi.

che oggi impone al Senato, o meglio, alla maggioranza, di accettare a scatola chiusa

in cui non si crede non è la fine del mondo. Questa è una delle materie che attendeva da tempo di essere riordinata e che non registrava necessità ed urgenza.

a determinare le politiche culturali delle fondazioni. È un principio di ordine costituzionale, me ne rendo conto, però non vorrei che fosse l'inizio di un pensiero lungo che finirà poi per attribuire le competenze, quindi i finanziamenti, delle fondazioni alle Regioni, con le differenze che conosciamo

Ho finito. Le 14 fondazioni sono un patrimonio nazionale, e il concorso delle Regioni non deve in alcun modo sbiadire e ledere questa loro caratteristica.

«dal vivo». Qui si sta parlando dello spettacolo in generale. Lo spettacolo dal vivo, nella terminologia antiquata e premediatica che ancora vige da noi, è una tipologia molto definita, il che significa circoscrivere questa norma. Fate voi, ma è una sciocchezza.

Vittoria *(PD)*. Signora Presidente, con questo emendamento proponiamo un richiamo puntuale alle previsioni del Titolo V della Costituzione ed un richiamo alla competenza concorrente che le Regioni hanno su questa materia. infatti inaccettabile, come sospettiamo che il Governo voglia fare, lasciare la responsabilità delle risorse per fondazioni, almeno per alcune di queste, interamente alle Regioni. Certamente, signor Ministro, questo testo che le Camere hanno hanno quasi approvato in prima e seconda lettura e che si accingono ad approvare in terza lettura in via definitiva è un po' meno cattivo di quello che il Governo ha proposto: un tantino meno cattivo. Comunque, secondo noi, la soluzione

Riforma vera, però, non un brutto decreto con delega, come ha proposto il Governo. Per questo stiamo contestando il provvedimento e siamo dispiaciuti che nessuno dei nostri emendamenti veri, come quelli che, per esempio, miravano alla defiscalizzazione dei contributi privati, sia stato accettato.

Senato non approva**.

ad approvare questo pessimo provvedimento, noi dell'Italia dei Valori desideriamo utilizzare questa nostra dichiarazione di voto per esprimere tutta la nostra solidarietà ai lavoratori del mondo dello spettacolo che ormai da anni vengono mortificati dalla vostra azione di governo.

desideriamo esprimere tutta la nostra solidarietà ai lavoratori del mondo dello spettacolo, che ormai da tempo vengono mortificati dalla vostra azione di governo. Abbiamo provato in tutti i modi e in entrambi i rami del Parlamento a farvi comprendere che ciò vi apprestavate a fare rappresentava un durissimo attacco alla cultura del nostro Paese e alla dignità dei lavoratori di tutto il mondo dello spettacolo. Da molto tempo le abbiamo offerto, signor Ministro, la nostra totale disponibilità a riprendere il percorso avviato dalla Commissione istruzione del Senato un anno fa ed individuato nella risoluzione, a firma

abbiamo quindi provato alla Camera dei deputati con i colleghi dell'Italia dei Valori per 40 ore di seguito, compresa la notte, a farvi comprendere la gravità di quello che stavate facendo. Oggi, in terza lettura al Senato, nei 20 minuti assegnati al nostro Gruppo - 20 soltanto! le nostre preoccupazioni e le nostre perplessità vengono confermate. Noi diciamo con forza "no" a questo provvedimento, lesivo della dignità dei lavoratori del mondo dello spettacolo, e alla mortificazione che oggi stanno subendo grazie alla vostra arroganza e alla vostra testardaggine; ci uniamo al grido di allarme che giunge da tutti i lavoratori delle fondazioni liriche italiane: dagli studenti dei conservatori e dalle loro famiglie, dagli artisti internazionali che invocano con forza la non approvazione di questo decreto. Tutto il Paese continua a lanciare appelli e a protestare contro questo iniquo decreto che umilia le professionalità teatrali, disincentiva la formazione e gli studi musicali, ma soprattutto mortifica la nostra stessa cultura. Ribadiamo Ribadiamo con forza che l'assenza di una vera strategia riformatrice ha portato il settore al collasso e gli interventi contenuti nel decreto prevedono soltanto forme repressive: non una parola, non una nuova idea, non un suggerimento per rilanciare il settore, ma soltanto repressione, tagli, licenziamenti e azzeramento di ciò che certamente ha bisogno di essere riformato. L'impostazione L'impostazione generale del decreto tende, infatti, ad identificare nel costo del personale il principale, se non unico, elemento di spreco di sistema, da correggere attraverso tagli che non sono frutto di una corretta revisione degli istituti contrattuali, ma solo intervento acritico e centralista di riduzione dei salari. Per noi dell'Italia dei Valori il personale rappresenta l'elemento più importante e imprescindibile per costruire il prodotto teatrale: l'opera lirica, i concerti sinfonici, i balletti, gli spettacoli di prosa non potrebbero aver luogo senza professori d'orchestra, artisti del coro, ballerini, tecnici, macchinisti, costruttori che costituiscono proprio quella voce di costo sulla quale il Governo intende intervenire con il decreto oggi in discussione. Forse lei, signor Ministro, non lo sa, ma per realizzare un'opera o un balletto bisogna disporre di centinaia di masse artistiche e tecniche professionalmente preparate, che devono essere considerate parte viva ed indispensabile della produzione, alla stregua degli interpreti vocali, del direttore d'orchestra, del regista, del coreografo, dello scenografo-costumista e di un corollario di altre importanti figure connesse alla sua realizzazione (questi ultimi professionisti esterni all'organizzazione ma per i quali, tuttavia, non si bada a spese). Il teatro lirico, infatti, è come una grande fucina dove convive un personale variegato e altamente specialistico in campo musicale (maestri, orchestra, coro e ballo) e tecnico (macchinisti, attrezzisti, elettricisti, scenografi, sarti, parrucchieri, truccatori) e al momento di andare in scena è necessario che tutto vada alla perfezione, che le professionalità siano esercitate al meglio e che i protagonisti dell'allestimento scenico e musicale siano all'altezza della situazione. pensare che si possa essere competitivi nella precarietà ed episodicità dell'offerta lavorativa è sicuramente aberrante. Non bisogna dimenticare che la stabilità ottenuta dal personale dei teatri non è solo una conquista sociale, ma è anche sinonimo di qualità artistica e professionale. Il problema, piuttosto, sta nella presunzione di chi si accosta a questo mondo senza conoscerlo a fondo. Solo chi vive la vita quotidiana di un teatro lirico può capire le problematiche che riguardano la messa in scena di uno spettacolo. Non è condivisibile, pertanto, non considerare il personale dei teatri lirici come spesa viva necessaria per la produzione. Varie tipologie di personale, costantemente coinvolte, che possono sembrare superflue a chi non conosce la materia, sono indispensabili per consentire alla fine la fruizione della spettacolo al pubblico.

Senza di essi il grande melodramma, che rappresenta da sempre uno dei prodotti più importanti dell'Italia nel mondo, non potrebbe ogni sera essere messo in scena in tutto il Paese, e alla fine l'Italia sarebbe più povera di quello che già è per effetto delle politiche culturali miopi del Governo. Ormai le politiche culturali del Governo sono chiare; dopo il massacro nella scuola, i cui tagli indiscriminati hanno creato tanta disoccupazione come mai si era mai vista nei settori che producono cultura, il disegno dello smantellamento culturale perseguito da questo Governo continua con le fondazioni liriche e i teatri. Signor Ministro, avrebbe fatto bene ad ascoltare il grido che si è levato dai grandi artisti che lavorano nei nostri teatri e che meglio di tutti noi conoscono la specificità del loro lavoro e la specificità del lavoro nelle nostre istituzioni musicali. Avrebbe fatto bene ad ascoltare almeno Carla Fracci, Zubin Mehta, Luca Ronconi. Luca Ronconi. Cosa dicono da mesi questi grandi artisti? Dicono che è importante la stabilità; è importante il far musica insieme; è importante crescere insieme come gruppo. Dicono che è importante selezionare i migliori talenti

di dare certezza almeno triennale all'intero comparto delle fondazioni, signor Ministro, non solo a quelle fondazioni cui il Governo avrebbe intenzione di conferire uno *status* di autonomia rispetto alle altre.

ci vuole competenza e volontà di fare. Noi la nostra disponibilità l'avevamo offerta, ma voi l'avete mortificata e calpestata. Con la vostra arroganza e schizofrenia state scrivendo una brutta pagina di storia, un durissimo attacco alla cultura italiana di cui dovete assumervi tutta la responsabilità davanti ad un Paese che vi guarda sbigottiti. Noi non ci stiamo e voteremo convintamente no al provvedimento in esame. Ci saremmo aspettati un atto di orgoglio

Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad approvare un provvedimento di grande interesse riguardante le fondazioni liriche, dopo che la Camera ne ha dibattuto nel corso di una maratona imposta dall'esigenza di licenziarlo in breve tempo, per permettere il definitivo avallo prima dell'imminente scadenza. I tempi contingentati, che in particolare alla Camera non hanno permesso l'opportuno approfondimento che noi auspicavamo, sono dovuti di certo alla stessa natura del decreto-legge quanto mai inopportuna in una materia così complessa, così implicante e così delicata. Per primi abbiamo riconosciuto l'opportunità di intervenire in questo settore della musica e degli enti lirici, denunciando il fallimento della legge Veltroni e sottolineando la mancanza della responsabilizzazione di una *governance* eccessivamente disinvolta nella gestione delle risorse, che ha condotto ad una situazione al limite del collasso, che avrebbe richiesto per tempo una decisiva sterzata ai fini di un drastico contenimento degli sprechi, attraverso l'ottimizzazione della gestione, la razionalizzazione della stessa *governance*, la valorizzazione delle eccellenze, a tutela soprattutto dei lavoratori che non avrebbero dovuto rispondere di scelte a cui non hanno concorso e che hanno portato alle conseguenze disastrose che sono sotto i nostri occhi. signor Ministro, pur consapevoli dell'esigenza di dover tempestivamente intervenire, abbiamo ritenuto sin da subito che il decreto-legge non fosse lo strumento più opportuno, *in primis* in quanto avrebbe compresso il necessario ampio confronto sul tema e in secondo luogo perché avrebbe condotto ad un intervento settoriale e affatto organico. Le nostre preoccupazioni purtroppo si sono rivelate fondate. Lo testimonia il rapido esame alla Camera che si è svolto con una vera e propria "maratona" e la nostra convocazione dettata dalla necessità di approvare il provvedimento modificato a ridosso della scadenza. Non è l'opportunità dell'intervento che critichiamo, ma il modo con cui viene fatto e per tre fondamentali ragioni, già espresse nelle argomentazioni delle pregiudiziali discusse nell'altro ramo del Parlamento. *In primis* l'esigenza di intervenire per il riordino di questo delicato settore, fondamentale anche per la competitività culturale del nostro Paese, c'è, nessuno la nega, ma questa è lungi dal poter essere scambiata *tout court* con i requisiti di necessità e di urgenza previsti in via straordinaria dalla Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Inoltre, lo stesso articolo 1, con cui si stabiliscono dei generici criteri di riordino, conferendo al Governo un'amplissima potestà di regolamentazione delegificante, è in contrasto con la natura del decreto-legge in quanto è escluso che si possa far ricorso alla decretazione d'urgenza se non per l'introduzione di norme di immediata applicazione di contenuto univoco ed omogeneo, nonché specifico. Vi è poi un intervento statale molto denso e molto esteso sulla stessa organizzazione delle fondazioni lirico-sirifoniche. Questo decreto-legge, infatti, a nostro avviso interviene a gamba tesa sull'autonomia delle fondazioni, conferendo un potere amplissimo al Governo sotto tutti i profili, con un'ottica statalista, in evidente contrasto con la dimensione federalista tanto sbandierata dalla maggioranza in mille occasioni, con la volontà soprattutto di adottare criteri manageriali e privatistici nella *governance* e nella gestione delle fondazioni stesse.

Dei passi in avanti sono stati fatti grazie soprattutto alle proposte dell'opposizione, in particolare a tutela dei diritti acquisiti dei lavoratori; mi riferisco allo spinoso tema del trattamento economico aggiuntivo, frutto della contrattazione integrativa. avremmo voluto che il Governo avesse mostrato maggiore coraggio e sensibilità verso un settore così importante per la cultura del nostro Paese. Al contrario, sembra che questo provvedimento si limiti ad individuare nel solo costo del personale l'unico elemento di spreco, mentre a nostro avviso bisognava *in primis* individuare le responsabilità di questa situazione emergenziale, per trovare poi le soluzioni, indicare una precisa *governance*, predisporre più stringenti controlli sulle gestioni, avviare concrete sinergie tra le fondazioni, predisporre una circuitazione delle produzioni stesse, valorizzare quelle eccellenze che ci sono e colmare i deficit culturali di alcune Regioni svantaggiate, prevedere infine *partnership* private. Tutto questo, purtroppo, nel provvedimento non c'è, perché ci si è limitati a tracciare ampi e generici criteri a cui dovrà attenersi il Governo in via regolamentare. Se noi condividiamo che una gestione improntata a criteri manageriali, unitamente all'innesto di risorse private, potrebbe essere la strada per una ripresa economica del settore, restiamo però perplessi di fronte alle deboli misure che vengono adottate per attrarre capitali privati a fronte di risorse pubbliche, che sono assolutamente esigue, signor Ministro, quali quelle stanziate con il Fondo unico per lo spettacolo.

Avremmo voluto ben altro. In primo luogo, avremmo voluto l'approvazione della legge sullo spettacolo dal vivo, che è all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento, intorno alla quale sembra essere maturato un ampio consenso. Con essa si sarebbe potuta creare quella cornice di carattere più ampio, nell'ambito della quale affrontare anche il tema più specifico delle fondazioni liriche. Ma così non è stato. Quindi, ci dobbiamo soltanto augurare che si possa fare di più e di meglio, portando a conclusione l'*iter* di approvazione del disegno di legge relativo alla riforma dello spettacolo dal vivo. L'impianto del provvedimento al nostro esame, infine, non è assolutamente soddisfacente, né può considerarsi una sufficiente garanzia per lo stesso comparto e i suoi addetti, alla luce dei numerosi attacchi che più volte purtroppo questo Governo, attraverso la figura del Ministro all'economia, ha sferrato nei confronti della cultura in svariati settori, attacchi parzialmente e qualche volta sventati anche grazie all'intervento del Capo dello Stato. Questo decreto-legge risulta ancora fortemente penalizzante e per nulla affatto riformatore nella misura in cui non prevede incentivi fiscali alla cultura, così come in Europa e dovunque è stato fatto. Al tempo stesso, riduce gli stanziamenti pubblici previsti dal Fondo unico per lo spettacolo. Non permette, una programmazione sulla base di risorse certe e, in assenza di risorse certe, non si può programmare neanche nel mondo e nello spazio della cultura. Costringe quindi le fondazioni all'esoso ricorso all'indebitamento, continua a promuovere la precarizzazione dei rapporti di lavoro, disconosce il ruolo dei professionisti dello spettacolo e della cultura.

maturate in anni e anni di sacrifici, da un mercato del lavoro mortificante, che non li rispetta prima di tutto nella loro dignità. Dignità significa sopratutto - signor Ministro, me lo lasci dire arrivare al riconoscimento previsto dalla legge n. 508 per quanto riguarda i diplomi rilasciati dai conservatori, che devono essere considerati diplomi di laurea, così come la stessa legge ha stabilito. Fino ad oggi, però, non abbiamo visto le conseguenze di questo dettato legislativo che ancora giace lì inerte e nessuno se ne occupa.

Questo è intollerabile e mortifica la loro stessa dignità e creatività. L'Italia possiede circa la metà del patrimonio artistico mondiale. L'economia basata sulla cultura, a cui naturalmente il nostro Paese è vocato e che ha sempre rappresentato un fetta importante del nostro sistema produttivo,

L'attenzione alla cultura ci permetterebbe di salvaguardare l'evoluzione, di scongiurare una deriva involutiva del nostro Paese e di essere più fedeli alla nostra stessa identità, che è assolutamente e prima di tutto di spirito e di cultura, difendendo una tradizione non elitaria

di un popolo, la sua consapevolezza democratica che vive di relazioni, di conoscenza, di interscambio e di cooperazione: tutti fattori di libertà che non possono essere compressi, pena la morte della creatività, che è il vero valore aggiunto del nostro Paese. Per tutte queste ragioni, non posso che esprimere, a nome del mio Gruppo, un voto contrario al provvedimento in Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il provvedimento sul quale ci apprestiamo ad esprimere il voto è frutto di un percorso lungo e articolato, a dimostrazione che nell'agenda politica la cultura occupa un ruolo non secondario. Le Camere, affermando con decisione la centralità del Parlamento, hanno affrontato le questioni in discussione in profondità e direi con risultati discreti, visto il momento di difficoltà generale per quanto riguarda l'economia. Ricordo che in questi anni le fondazioni lirico-sinfoniche non sono riuscite a gestire in modo ottimale la loro natura di soggetti di diritto privato, disperdendo forze ed energie. Si è reso urgente un provvedimento che affrontasse i gravi problemi gestionali delle fondazioni. Parliamo di perdite per 200 milioni di euro e interessi passivi per 9 milioni e mezzo di euro. Le fondazioni hanno accumulato debiti per 300 milioni di euro. Compito e responsabilità del Governo era di intervenire con urgenza in un settore che assorbe quasi il 50 per cento del Fondo unico per lo spettacolo e che a tutt'oggi è finanziato solo per il 20 per cento dagli investimenti privati e dai ricavi dei biglietti, e per il restante 80 per cento dai fondi pubblici. Un settore che presenta costi straordinariamente elevati rispetto ai profitti. Il decreto presentato inizialmente dal ministro Bondi è stato modificato grazie agli importanti contributi emendativi dei diversi Gruppi parlamentari. Il nostro, in particolare, all'articolo 1 ripropone buona parte delle indicazioni presenti nella risoluzione approvata in Commissione cultura all'unanimità il 18 marzo 2009. Proposte atte a favorire una maggiore stabilità del settore, rispondendo al principio dell'intervento culturale come investimento e non come spesa. Una linea che come Lega Nord ci porta a esprimere voto favorevole a questo provvedimento. Presidente, signor Ministro, colleghi, a nome del Gruppo del Partito Democratico esprimo con profonda amarezza un voto contrario a questo provvedimento, stonato e votato, purtroppo, nell'indifferenza

Siamo ormai al sessantesimo decreto-legge di questa legislatura: una misura eccezionale utilizzata come strumento ordinario, che, mentre altrove si parla o si straparla di federalismo e si tagliano risorse a Regioni ed enti locali, tocca in modo evidente la ripartizione di competenze fra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già preannunciato che impugneranno il decreto. Ma soprattutto, neppure gli scioperi e le rappresentazioni annullate negli ultimi giorni nei teatri più importanti del nostro Paese, conosciuti in tutto il mondo, hanno portato il minimo ravvedimento nel Governo in nome del fatto che il nostro Paese è conosciuto nel mondo anche e specialmente per la lirica, il teatro, la danza, il balletto. Nel marzo 2009 la 7a Commissione del Senato, all'unanimità, con il consenso del Ministro, aveva approvato una risoluzione

in cui si invitava il Governo ad aumentare le risorse del FUS, a favorire una maggiore stabilità del settore tramite gli strumenti di finanziamento a carattere pluriennale, a disciplinare con chiarezza negli statuti i compiti dei vari organi, con l'impegno a costruire insieme in tempi determinati un disegno di legge condiviso. Questo percorso serio e responsabile è stato abbandonato con una decretazione d'urgenza giustificata anche recentemente dal Ministro in quest'Aula con l'esigenza di evitare il fallimento del settore, ma l'unica verità è che si condanna la quasi totalità dei nostri teatri al declassamento, e qualcuno alla chiusura. Come si fa, infatti, ad aiutare le nostre fondazioni liriche tagliando le risorse pubbliche e votando contro i nostri emendamenti che miravano a favorire la defiscalizzazione dei contributi dalle imprese dei privati? Basterebbe leggere i bilanci delle fondazioni per capire che uno dei nodi irrisolti è la scarsa partecipazione dei privati. Era questo il senso vero delle fondazioni, ovvero uno strumento idoneo ad attirare capitali privati, oltre che il sostegno delle amministrazioni locali, fermo restando un fondamentale coinvolgimento statale. Eppure ne esistevano di percorsi alternativi. Basti pensare al disegno di legge n. 1256, presentato nella scorsa legislatura dall'allora senatore Fontana, che introduceva criteri di premialità rispetto al merito e che maggioranza e opposizione decisero congiuntamente di firmare. Il Partito Democratico, che lei giustamente ha prima evocato, insieme al resto dell'opposizione ha ottenuto miglioramenti al testo sia al Senato che alla Camera, come ad esempio lo stralcio dell'articolo 5, e ne rivendica tutti i meriti. Il Partito Democratico non può però accettare, signor Ministro, che questo provvedimento non sia che l'ultimo in cui lei assiste passivamente al saccheggio delle risorse sulla cultura italiana, mentre nella manovra economica si provvede a sciogliere d'ufficio l'Ente teatrale italiano e a tagliare della metà i contributi, già esigui, agli enti culturali. Mi consenta, ministro Bondi, una citazione manzoniana benevola, che, per evitare malintesi tra noi, vista anche la stima che le porto, è riferita al provvedimento e non certo alla sua persona. Anche donna Prassede era convinta di adoperarsi al bene di Lucia, ma, come sottolinea Manzoni, aveva poche idee, di cui la gran parte confuse, e non erano di quelle che le erano meno care. È il ritratto di questo provvedimento: poche idee, la gran parte confuse e che - ho l'impressione - sono quelle che le sono più care. Così, nonostante la crisi, non avvengono le stesse scelte politiche per il sapere e la cultura in altri Paesi europei come, ad esempio, in Francia e in Germania.

quella tradizione culturale a cui dobbiamo prestigio, riconoscenza e gratitudine e per la quale il nostro Paese è conosciuto nel mondo. Il decreto oggi in votazione di sicuro non sarà ricordato per questo. Signor Presidente, signor Ministro, care colleghe e cari colleghi, sul provvedimento alla nostra attenzione in prima lettura il 16 giugno scorso il Senato ha già espresso un netto voto favorevole con la piena adesione del Popolo della Libertà. Il provvedimento ritorna ora al nostro esame modificato alla Camera dei deputati in una decina di punti. Si tratta di modifiche minori e assolutamente condivisibili, che portano a ribadire sul provvedimento in esame il convinto voto favorevole del Popolo della Libertà. Sulle modifiche apportate dalla Camera consentitemi, tuttavia, due osservazioni che faccio anche in relazione al recente intervento del senatore Procacci. Quanto alla prima osservazione, all'articolo 1, comma 1, tra i criteri cui dovrà attenersi il Governo nella formulazione del regolamento o dei regolamenti di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle fondazioni lirico-sinfoniche, la Camera dei deputati ha aggiunto, tra gli altri, il criterio f‑*bis)*. Questo criterio postula l'individuazione delle modalità con cui le Regioni devono concorrere, secondo le proprie competenze, a supporto dello spettacolo dal vivo. Le fondazioni lirico‑sinfoniche sono certamente una forma di spettacolo dal vivo, ma il criterio f‑*bis)*, se pretende di allargare il compito dei suddetti regolamenti a tutto il settore dello spettacolo dal vivo, deborda nettamente dall'ambito della delegificazione disposta dall'articolo 1. Seconda osservazione. Un emendamento approvato alla Camera al comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che, nel caso in cui non si riesca a stipulare entro i prossimi due anni un contratto collettivo nazionale di lavoro, «eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti». La formulazione tende a nascondere il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche che non avranno ancora raggiunto a fine biennio il pareggio del bilancio, del diritto a conservare gli eventuali trattamenti economici aggiuntivi previsti. Tornando alle valutazioni complessive sul provvedimento in esame, ne ribadiamo gli aspetti molto positivi già sottolineati nella dichiarazione di voto del 16 giugno. Alla base vi è la profonda convinzione che l'opera lirica e la musica sinfonica costituiscono ricchezze culturali di grandissimo pregio, componenti fondamentali del patrimonio identitario del nostro Paese, sia nella percezione di noi cittadini italiani, sia nella percezione dei cittadini di tanti Paesi esteri. Alla base vi è anche la piena consapevolezza dell'eccezionale ruolo svolto dalle fondazioni lirico-sinfoniche nel "ri-creare" prodotti culturali di straordinario valore, nel diffondere cultura teatrale e musicale di alta qualità, nel rivivificare le nostre grandi tradizioni musicali. È proprio tale consapevolezza, unita alla viva preoccupazione per le difficili e precarie condizioni economiche del settore, ad aver determinato il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare il provvedimento d'urgenza del decreto-legge alla nostra attenzione.

L'articolo 1 prevede una delegificazione del settore, con l'affidamento al Governo della revisione dell'attuale loro assetto ordinamentale ed organizzativo, da attuare su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, tramite uno o più regolamenti emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L'articolo 2 definisce come sarà formata la delegazione rappresentativa per la parte datoriale delle fondazioni lirico-sinfoniche che discuterà e sottoscriverà il contratto collettivo nazionale di lavoro. L'articolo 3 contiene varie disposizioni in materia di personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, riguardanti assunzioni, prestazioni di lavoro autonomo, stipulazione di contratti integrativi al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, trattamento economico per le missioni all'estero, nonché la fissazione dell'età anagrafica di 45 anni per la nuova età pensionabile delle ballerine e dei ballerini. Dei successivi articoli meritano di essere menzionati, in particolare, l'articolo 7, che prevede una serie di disposizioni per l'avviamento della nuova IMAIE (Istituto mutualistico per la tutela degli artisti autori che ne garantiranno il buon funzionamento, e l'articolo 7-*bis*, aggiunto durante l'esame al Senato, che istituisce la festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, il giorno 17 marzo 2011. Sull'argomento delle fondazioni lirico-sinfoniche, come ha ribadito poco fa anche il Ministro, le forze politiche hanno dimostrato nel dibattito parlamentare di condividere molti punti. Valutazioni condivise, oltre a quella del grande valore culturale delle fondazioni lirico-sinfoniche nella vita del nostro Paese, sono, ad esempio, il pieno riconoscimento della natura pubblico-privata delle fondazioni; la preoccupazione per le attuali gravi difficoltà economiche del settore; la consapevolezza dell'urgente necessità di un intervento legislativo volto a far recuperare condizioni di serenità finanziaria; la necessità di imprimere un forte impulso imprenditoriale alla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche per garantire rispetto dei vincoli di bilancio e adeguata promozione della produttività; la consapevolezza della necessità di un forte ridimensionamento dei contratti integrativi stipulati a livello delle singole fondazioni, spesso presentanti degenerazioni corporative, a favore di un pieno recupero dell'importanza del contratto collettivo nazionale di lavoro. Di fronte a questa estesa condivisione di elementi primari della questione delle fondazioni lirico-sinfoniche, è singolare che durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge del Governo, sia al Senato sia alla Camera dei deputati, vi sia stato invece un contrasto politico assai aspro. Alla Camera, per riuscire ad approvare il provvedimento in Aula nonostante l'opposizione ostruzionistica dell'Italia dei Valori, vi è stata la necessità di una seduta fiume, iniziata alle ore 10 di mercoledì 23 giugno e terminata, senza interruzioni, giovedì 24 giugno, alle Non riesco francamente a comprendere le ragioni di tanta asprezza e, signor Presidente, sono personalmente dell'avviso che l'utilizzo di tecniche ostruzionistiche in questa circostanza non trovi assolutamente giustificazioni e costituisca un uso gravemente distorto dei Regolamenti. Concludo la mia dichiarazione di voto, signor Presidente, rivolgendomi a lei e chiedendole un'attenta considerazione dell'opportunità di modificare il Regolamento del Senato, sia per le attività in Commissione sia per le attività in Aula, onde evitare che si ripetano vicende parlamentari simili a quella sperimentata per questo provvedimento, onde consentire cioè che in parallelo alla indispensabile tutela dei diritti delle minoranze vi sia anche piena tutela dei diritti di decisione della maggioranza, nel rispetto del voto dei cittadini.

Come lei saprà, da alcune settimane la Commissione affari costituzionali è impegnata nell'esame del disegno di legge n. 2180, a prima firma del senatore Gasparri.

per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i Ministri, consistenti nella sospensione dei processi. *(Brusìo).*

immunità, una nuova prerogativa immunitaria per le alte cariche dello Stato successivamente alla fase in cui viene esercitata l'azione penale: è il cosiddetto lodo Alfano costituzionalizzato. La Commissione affari costituzionali sta svolgendo

ma anche perché il valore di rango costituzionale delle norme che si stanno discutendo pretenderà un domani l'interpretazione delle disposizioni - qualora venissero approvate dal Parlamento - anche alla luce del criterio ermeneutico della volontà del legislatore. Sarebbe quindi molto utile, sia per la pienezza delle informazioni, sia per la ricostruzione del criterio interpretativo della volontà del legislatore, poter disporre di

gli Uffici mi dicono che questa stessa regola è stata seguita nelle occasioni in cui, nelle legislature precedenti, il Senato si è occupato di riforme costituzionali.

È nella facoltà del Presidente compiere una valutazione, al di là di questi precedenti, di quanto il Regolamento stesso prevede. Farò presente questa sua richiesta al presidente Schifani. **Per un sollecito

Presidente, utilizzerò al meglio questa giornata, per noi romani, festiva, che immagino avrà delle analogie quando si tratterà di Sant'Ambrogio, Santa Rosalia e così via.

ha redatto un testo unico in circa sei o sette mesi dall'inizio della legislatura; dopo di che siamo stati presi in ostaggio, come ormai accade a tutti in quest'Aula, dalla Commissione bilancio. Evidentemente funziona il medesimo meccanismo della logica politica del saldo invariato, che sarebbe la fine della politica, se volessimo discuterne, perché la politica è priorità di scelta. è ormai più di un anno che il testo unificato è stato consegnato alla 5a Commissione per l'espressione del relativo parere. Non siamo solo d'accordo noi di maggioranza e opposizione, ma perfino il sottosegretario Mantovano è venuto due volte a sollecitare il provvedimento. Poiché è un disegno di legge condiviso, poiché il caso di Elisa Claps ha riportato tristemente alla luce questo tema, poiché è un tema su cui finalmente far bella figura con i cittadini

sono uscite. Si può dire che finché non c'è comunicazione ufficiale il Governo non può dire niente e il Parlamento non può chiedere. Però qui siamo al paradosso che la comunicazione ufficiale non c'è, ma che un ministro della Repubblica, il ministro Calderoli, rilascia un'intervista al "Corriere della Sera" in cui dà quattro spiegazioni su cosa dovrebbe fare Brancher: primo, sarebbe stato un ottimo ministro dell'agricoltura;

l'abbiamo conosciuto perché è venuto in Commissione a parlarci di federalismo in Germania, in particolare nella Bassa Sassonia: non so se è prevista una delega su questo o se magari gli verrà data la delega sul lodo Alfano costituzionale, con cui risolverebbe il problema dell'impedimento. Però non è ammissibile che il Ministro ci chieda di giudicarlo sulla base delle deleghe

si è addirittura consumato un suicidio in una camera di sicurezza. Oggi i reclusi dell'Ucciardone, con tragica ironia, scrivono in una lettera inviata all'ufficio del Garante dei detenuti e alla stampa che forse per svuotare le carceri si attendono altri suicidi. Giovedì in molte carceri cominceranno azioni di civile protesta.

L'incremento di reclusi nelle carceri italiane oscilla tra le 500 e le 700 unità al mese: moltiplicate questa cifra per cinque anni, sommatela ai 68.000 reclusi che in questo momento si trovano nelle carceri nelle carceri italiane e facilmente comprenderete, alla luce delle suddette cifre, quanto sia drammatico il problema. Allora, va bene portare avanti iniziative che prevedano pene alternative nell'ultimo anno di detenzione, ma anche in quel caso bisogna capire come scrivere le norme, altrimenti si rischia di risolvere un problema e di crearne altri cento o di non risolvere affatto il problema del sovraffollamento. Credo sia irrinunciabile

all'adeguamento dell'organico della polizia penitenziaria (abbondantemente al di sotto delle necessità) degli educatori e degli psicologi;

sortirebbe un effetto maggiore; mi riferisco alla commutazione in pene alternative diverse dalla detenzione per i reati di minore allarme sociale o che comunque non siamo atti di violenza. Sulla base di questa premessa, signor Presidente, mi permetto di chiederle di sollecitare al Ministro della giustizia la risposta a tutte le interrogazioni che portano la firma del sottoscritto e che riguardano complessivamente le condizioni delle carceri.

Passo piuttosto a trattare un tema completamente diverso. Sono qui a sollecitare la risposta ad una serie di interrogazioni che riguardano grosse strutture sanitarie della città di Roma e della Regione Lazio. In questi ultimi quindici giorni i direttori generali uscenti hanno monopolizzato l'intero bilancio di questi enti con promozioni

che per accontentare gli amici degli amici imporrà alla Regione Lazio per i prossimi cinque anni di subire contratti fatti non si sa a chi e non si sa perché. Faccio un esempio, Presidente, e concludo. Queste grosse strutture sanitarie, e in generale la sanità del Lazio e di altre quattro Regioni, sono sotto commissariamento.

prendo atto delle sue considerazioni. È vero che si tratta di una Regione sottoposta ad una forma di commissariamento e quindi ci sono responsabilità come quelle che lei diceva; pertanto, nel dare